l'ANAS ha indicato le previsioni di intervento a breve termine per ridurre i disagi alla circolazione e successivamente la descrizione degli interventi programmati.

e procedono come da cronoprogramma. Per consentire i lavori del cantiere sito al chilometro 178+700 (svincolo San Piero in Bagno) della carreggiata sud della SS 3 *bis* Tiberina, è stato necessario chiudere al traffico della carreggiata sud e deviare il traffico sulla carreggiata nord con doppio senso di circolazione. Si illustra di seguito la situazione aggiornata della circolazione veicolare in transito lungo la SS 3 *bis* Tiberina nel tratto Verghereto-Bagno di Romagna, ove sono in corso i lavori di adeguamento al tipo IIICNR/80 con le seguenti limitazioni/deviazioni di carreggiata: chiusura della carreggiata nord (direzione Ravenna) tra il chilometro 177+300 e la conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta tra le medesime progressive; chiusura dell'ingresso in SS 3 *bis*, per il traffico che proceda in direzione Ravenna, dello svincolo di San Piero in Bagno al chilometro chiusura della corsia di marcia della carreggiata sud (direzione Roma) tra il chilometro 175+800 e il chilometro 177+300; chiusura della corsia di sorpasso della carreggiata nord (direzione Ravenna) tra il chilometro 175+800 chiusura della carreggiata sud (direzione Roma) tra il chilometro 175+750 ed il chilometro 175+820 e la conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta tra le medesime progressive. Disciplina questa prevista sino al 30 giugno 2010 come da ordinanze. Il tratto emiliano di statale risulta essere attualmente soggetto alle ulteriori deviazioni/limitazioni dovute alla presenza dei rispettivi cantieri dei lavori di manutenzione straordinaria,

del viadotto Case Bruciate posto tra il chilometro 170+359 ed il chilometro 172+200 è stata prevista la deviazione del traffico veicolare che proceda in direzione Roma, tra il chilometro 172+450 (bretella di uscita provvisoria - località Bagno di Romagna) ed il chilometro 168+200 (svincolo di Verghereto) sulla SP 137. È inoltre disposta la chiusura della corsia di sorpasso in carreggiata Nord (direzione Ravenna) tra il chilometro 170+200 e il chilometro 172+250, prevista sino al 10 marzo 2010 come da ordinanze. Per la presenza di lavori di miglioramento statico e del livello di servizio del viadotto Fornello, sito al chilometro 167+800 (località Verghereto), è stata disposta la chiusura al traffico della carreggiata Sud (direzione Roma) e conseguente istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, in carreggiata opposta (carreggiata direzione Ravenna), in corrispondenza del viadotto Fornello al chilometro (transito a senso unico alternato tra il chilometro 167+900 ed il chilometro 167+000) prevista sino a tutto il 2010. Si ribadisce che i percorsi alternativi, in caso di limitazioni della circolazione sulla strada statale 3 *bis*, sono regolarmente concordati con gli enti locali gestori della viabilità secondaria; pertanto la lunghezza degli stessi e i disagi all'utenza sono spesso conseguenti alle limitazioni imposte dai Comuni nell'attraversamento dei centri abitati. In merito alla realizzazione del collegamento Orte-Mestre mediante finanza di progetto, si informa che è in corso la procedura VIA sul progetto preliminare.

Sottosegretario,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accertamento delle eventuali responsabilità degli amministratori del Comune di Gallipoli nella fase di approvazione, collaudo e successiva gestione del progetto per la realizzazione del mercato ittico, non rientra tra le competenze del Ministero dell'interno. Ciò soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha collocato le autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione. Pertanto, l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso gli atti di governo locale e le determinazioni che adottano, in merito alle quali non sussiste alcuna funzione di controllo, né di intervento dello Stato. Ciò non toglie che la vita delle amministrazioni locali, tanto più in particolari contesti territoriali, venga seguita con particolare attenzione dagli uffici dal Ministero dell'interno che, ove si concretizzino fattispecie di propria competenza per reiterate violazioni di legge, ovvero per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, non manca di attivare i necessari controlli sugli organi. Venendo ora alla vicenda segnalata dall'interrogante, dalla ricostruzione operata dalla prefettura di Lecce, emerge che i lavori di costruzione della struttura da destinare a mercato ittico all'ingrosso di Gallipoli sono stati completati verso la fine del 2003. Attualmente sono in corso le verifiche relative all'adeguamento degli impianti, in particolare quello elettrico, alla normativa vigente. Secondo quanto riferito dal responsabile comunale, al termine di tale attività sarà possibile avere un quadro puntuale dei lavori necessari per rendere funzionale e utilizzabile la struttura. Nel tempo l'area, rimasta inutilizzata, è stata effettivamente oggetto di occasionali tentativi di occupazione e si è fortemente deteriorata per incuria e assenza di manutenzione. Nel 2008 l'amministrazione comunale, decisa a recuperare l'intero complesso, ha chiesto alla Regione Puglia un finanziamento di 350.000 euro, che sono stati successivamente stanziati. Tali fondi, tuttavia, sono ritenuti insufficienti. L'amministrazione comunale, infatti, ha stimato che per il completamento dell'opera sarà necessario un ulteriore finanziamento di circa 150.000 euro. Quanto alle preoccupazioni di possibili connessioni tra la vicenda e la criminalità locale, la prefettura di Lecce ha comunicato che, allo stato, non sussistono elementi da cui si possano ragionevolmente profilare, nei confronti dell'amministrazione comunale di Gallipoli, responsabilità in ordine ad un possibile nesso tra la mancata realizzazione del mercato ittico e le endogene attività criminali. Nello spirito di collaborazione istituzionale che impronta i rapporti tra il Ministero dell'interno e gli enti pubblici territoriali, non si mancherà di svolgere opera di sensibilizzazione tramite la prefettura di Lecce per la risoluzione del problema segnalato dall'interrogante.

a questa mia interrogazione, presentata esattamente 13 mesi fa. Devo ritenermi comunque insoddisfatto di quanto ha appena dichiarato, soprattutto in relazione al primo quesito, quesito, quello di cui ha parlato anche lei. Non a caso, avevo voluto attirare la vostra attenzione e sollecitare un vostro interessamento su eventuali connessioni fattuali e temporali tra la mancata realizzazione del mercato ittico di Gallipoli e le attività criminali in corso nel territorio di riferimento.

- ancora una volta, voglio sottolinearlo, grazie alle intercettazioni telefoniche svolte dai Ros dei Carabinieri e dal Gico della Guardia di finanza Gallipoli è sotto indagine; nel registro degli indagati ci sarebbero in tutto 46 nomi di politici gallipolini, sia di destra, sia di sinistra ed i reati in questione sarebbero corruzione, concussione e turbativa d'asta. Come vede, quindi, onorevole Sottosegretario, eravamo sospettosi circa la questione della mancata realizzazione del mercato ittico, ma a quanto pare l'intreccio di interessi e rapporti tra esponenti politici e della malavita gallipolini, oggetto in queste settimane dell'analisi della procura e della prefettura, è molto più ampio di quanto temessimo. Mi meraviglia però la risposta che le ha fornito il prefetto Tafaro. A tal proposito, infatti, vorrei ricordare che il 9 giugno di quest'anno ho presentato un'altra interrogazione per segnalare un deprecabile episodio verificatosi il 23 maggio 2009 a danno dell'avvocato Tommaso Scigliuzzo. L'avvocato era candidato al Consiglio provinciale di Lecce per la lista Italia dei Valori e tra i vari temi di un suo comizio elettorale a Gallipoli aveva affrontato quello dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti in quel Comune, non mancando di denunciare procedimenti sospetti nella gestione del servizio. Come conseguenza di ciò, al termine del comizio, l'avvocato Scigliuzzo subì pesanti minacce da parte di due giovani secondo i quali non doveva più permettersi di «fare i nomi o di parlare di certe cose». sotto la lente della procura e della prefettura ci sono le elezioni comunali gallipoline dell'anno scorso e quelle provinciali della scorsa primavera. Come vede, signor Sottosegretario, a più riprese, noi dell'Italia dei Valori abbiamo sollecitato un vostro intervento che chiedo oggi al Governo ancora una volta, approfittando della sua presenza qui, affinché si scavi a fondo nelle vicende dell'amministrazione di Gallipoli, anche valutando l'opportunità di sciogliere, laddove possibile, il Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, come già successo all'inizio degli anni '90 - per cui Gallipoli è recidiva - scongiurando così, spero, il perpetrarsi di quanto è successo già al Comune di Fondi.

Mi riferisco all'interrogazione del senatore Lumia con la quale chiede informazioni in merito alla cessione da parte di Cinecittà Holding Spa, ora Cinecittà Luce Spa, dell'intera partecipazione nella società Mediaport. A tal proposito occorre ripercorrere le fasi della vicenda risultanti dagli atti della Direzione generale per il cinema, che esercita la vigilanza su Cinecittà, in modo da poterla rappresentare con la massima chiarezza. L'intervento di Cinecittà Holding Spa nel settore dell'esercizio cinematografico previsto dall'articolo 5-*bis* della legge n. 202 del 1993 era prevalentemente immaginato come forma di sostegno della cinematografia italiana ed europea così come risulta anche dai primi atti di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali con i quali è stata data applicazione alla suddetta norma. Cinecittà Holding, conseguentemente, è divenuta titolare del 100 per cento di un gruppo di società, il cosiddetto gruppo Mediaport, a partire da settembre 2003. Successivamente, l'intero settore dell'esercizio cinematografico ha conosciuto una obiettiva contrazione di mercato ed il gruppo Mediaport, al pari di tutti i più importanti operatori italiani ed europei, si è trovato ad operare in un settore generalmente in perdita. Nel periodo 2003-2006, ovvero nel ciclo triennale di *start-up*, il gruppo Mediaport ha prodotto risultati gestionali fortemente negativi in linea con gli andamenti medi generali di settore. Tutto ciò ha formato oggetto di attenzione sia da parte della Corte dei conti sia del Ministero dell'economia e delle finanze; quest'ultimo, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2006 di Cinecittà Holding, ha raccomandato di procedere ad una accelerazione nella dismissione della partecipazione in Mediaport al fine di evitare che il protrarsi di tale procedura potesse generare ulteriori conseguenze negative di carattere economico e patrimoniale. Sulla base dei nuovi atti di indirizzo, in particolare del 27 giugno 2006, Cinecittà Holding ha provveduto, attraverso una procedura competitiva, a selezionare un *advisor* di levatura internazionale con incarico di assistere la società nelle scelte di incremento dell'efficienza e/o della valorizzazione del gruppo Mediaport ovvero di una sua dismissione. L'analisi effettuata ha evidenziato che la soluzione più efficiente sarebbe stata la vendita in blocco o, in alternativa, seppure meno conveniente, la vendita parziale di alcuni siti. Sulla base di ciò, nei primi mesi del 2007, Cinecittà ha avviato una procedura per la selezione di un potenziale acquirente di Mediaport con esito di "gara deserta". Nel frattempo, la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) nel prevedere un regime particolarmente stringente circa la detenzione da parte delle pubbliche amministrazioni di partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha rafforzato l'esigenza di dismettere la partecipazione in argomento; tale previsione normativa è stata successivamente recepita nell'atto di indirizzo del Ministro del 6 giugno 2008. Cinecittà Holding, pertanto, ha avviato ogni possibile contatto al fine di addivenire ad una vendita in blocco ovvero a vendite frazionate e, nel corso della seconda metà del 2008, la società Farvem Real Estate S.r.l. ha manifestato la disponibilità ad acquisire l'intero gruppo Mediaport. La trattativa si è conclusa il 28 novembre 2008 con la vendita del gruppo e la formalizzazione di un'offerta obiettivamente conveniente per Cinecittà Holding, tenuto conto del fatto che la società acquirente ha riconosciuto a Cinecittà un prezzo di euro 100.000 all'atto del trasferimento; ha acquisito l'intero pacchetto societario del gruppo Mediaport; ha rilevato l'intero indebitamento pari ad euro 26,5 milioni, così come risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento alla data del trasferimento; ha contrattualmente garantito la continuità aziendale per almeno tre anni; contrattualmente garantito la valorizzazione delle unità aziendali ed il mancato ricorso a procedure di mobilità e/o licenziamenti collettivi per un periodo di almeno 36 mesi. Voglio peraltro segnalare, per completezza di informazione, che la società Globalplex, presentatrice dell'esposto citato dall'interrogante, nel corso del 2007, all'esito della citata procedura per la selezione di un potenziale acquirente, presentò una propria proposta per rilevare tre dei nove siti del circuito in argomento. La proposta della Globalplex prevedeva, peraltro, il trasferimento dei predetti tre siti comprensivi di un immobile di proprietà del valore di circa 7 milioni di euro nonché l'esclusione di ogni debito residuo destinato a restare in carico a Cinecittà Holding, a fronte del pagamento di un prezzo di 2 milioni di euro. La predetta proposta, peraltro non formalizzata in forma vincolante, avrebbe comportato una perdita di bilancio per Cinecittà Holding, solo sui citati tre siti, di oltre 14 milioni di euro. L'offerta Globalplex quindi risultava estremamente più svantaggiosa, oltre che parziale, rispetto a quella presentata dalla Farvem Real Estate. Sulla base di quanto esposto, evidenzio che la procedura di dismissione risulta essere stata condotta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto delle procedure sindacali, pur formalmente non necessarie nel caso specifico, con esito di integrale apprezzamento da parte delle organizzazioni sindacali. Ciò tenuto conto anche della circostanza che gli stessi sindacati avevano espressamente fatto richiesta di una cessione in blocco del circuito al fine di una migliore tutela dei livelli occupazionali. Faccio inoltre presente che ogni singolo atto o decisione inerente la vicenda Mediaport è stato sottoposto all'attenzione del delegato della Corte dei conti, presente per legge in seno al Consiglio di amministrazione di Cinecittà; trasmesso, per opportuna informativa, alla vigilanza di questo Ministero che, proprio sulla base dei richiamati atti di indirizzo, ha costantemente monitorato le attività di Cinecittà Holding al fine di una celere e positiva risoluzione della vicenda. Con riferimento, infine, alle specifiche richieste del senatore Lumia, voglio evidenziare che Cinecittà Holding, al di là delle garanzie contrattuali, tutte ottenute, non può intervenire, né ovviamente può rispondere, delle scelte gestionali compiute dalla Farvem Real Estate

Presidente, non mi ritengo soddisfatto delle risposte fornite dal sottosegretario Nell'interrogazione avevo formulato, in modo chiaro, netto ed esplicito, due quesiti a cui il Sottosegretario non ha dato alcuna risposta. Il primo se i Ministri in indirizzo, all'atto della vendita, avessero preso tutte le misure necessarie per garantire la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali. Il secondo è se il Governo intenda il Governo intenda convocare un tavolo di confronto per discutere insieme alle organizzazioni sindacali e alla società Mediaport le preoccupazioni del mondo del lavoro e delle organizzazioni sindacali sul futuro dell'azienda e dei posti di lavoro, al fine di trovare soluzioni di garanzia in coerenza con la vendita che era stata fatta. lei ha ricostruito il percorso di dismissione, ma vorrei che verificasse meglio un punto che a me risulta diverso da quello che lei ha presentato, che riguarda l'indebitamente prodotto da Mediaport. A me risulta infatti che questo sia di 38,8 milioni di euro - quindi, un disavanzo ben più grande di quello che lei ha presentato e che solo 26,5 milioni di euro siano stati trasferiti al compratore, mentre i restanti 12 milioni sono rimasti a carico del venditore, cioè della società pubblica che lei qui ha richiamato, la Cinecittà Holding.

sulla continuità aziendale e occupazionale da garantire nei primi tre anni. Sono trascorsi solo pochi mesi e questi due punti sono venuti meno sono venuti meno perché già sul piano della continuità aziendale si sono avute dismissioni che contrastano con il principio iniziale, che era quello della vendita in blocco e non solo di alcuni siti.

anche delle prese di posizione da parte delle organizzazioni sindacali. Si registrano l'incombenza di sfratti esecutivi da parte degli affittuari delle sedi, problemi di pagamento con diversi fornitori e la scarsa manutenzione delle stesse strutture. Quindi, si è voluta fare una scelta - si può discutere se sia giusta o sbagliata - per rafforzare questo circuito, per affidarlo nelle mani solide di privati in grado di rilanciare e quindi di migliorare il tipo di investimenti che sono necessari a causa anche della trasformazione del mercato delle sale e delle novità che nel frattempo sono intervenute in questo settore. Di tutto ciò non abbiamo segnali,

che erano decisive, importanti, date a garanzia di una dismissione intelligente da parte del settore pubblico. Tutto ciò non è stato fatto; può recuperare, mi auguro che lo faccia, perché ripresenterò questa interrogazione, affinché vi sia da parte del Governo

dal custode giudiziario e liquidatore. Non vorrei che anche in quel caso si riproducessero, naturalmente in un contesto diverso da quello precedente, le stesse condizioni: prima una disponibilità all'acquisto e poi successivamente una cattiva gestione gestione e quella inefficienza che lei denunciava prima quando era in gestione da parte del settore pubblico. Signor Sottosegretario, ci ritorneremo,e la prossima volta mi auguro che arrivi pronto e puntuale sui punti che l'interrogante ha chiesto, e ritornerà a chiedere.

mi riferisco all'interrogazione della senatrice Germontani con la quale la stessa chiede informazioni circa le iniziative del Ministero per i beni e le attività culturali a salvaguardia dell'integrità di piazzale Berzieri e del complesso monumentale liberty-déco delle Terme Berzieri, bene già sottoposto a tutela con decreto del Ministro del 15 novembre 1993. A tale proposito rappresento anzitutto che l'attuale progetto di riqualificazione del piazzale e delle aree di pertinenze delle terme è maturato a seguito di numerosi incontri che si sono svolti tra i progettisti, il Comune e la locale sovrintendenza per individuare una soluzione di equilibrio volta a contemperare l'esigenza di tutela storica delle terme con la necessità di migliorarne la fruizione e la valorizzazione, attraverso progettazione di una piazza sul fronte principale in sostituzione di uno spazio di risulta caratterizzato esclusivamente dal traffico a ridosso dell'ingresso delle terme. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali di dettaglio e sulla base degli elementi di informazione forniti dagli uffici territoriali di questo Dicastero, faccio presente che sulla base del progetto originario degli architetti Bernardini e Giusti, mai attuato, la facciata dell'edificio termale avrebbe dovuto vedere il suo completamento con la sistemazione degli spazi esterni mediante rampe di accesso, a forma di esedra e aiuole, il tutto posizionato in asse all'ingresso principale. Di fatto la descritta sistemazione esterna non fu mai realizzata a causa di cedimenti del terreno. Pertanto, al tombinamento del torrente Citronia non non ha mai fatto seguito alcuna particolare sistemazione urbana di qualità per questo spazio a forma irregolare contraddistinto, da una parte, dall'importante facciata del palazzo Berzieri e, dall'altra, dal Pozzo Scotti, realizzato con cemento con cemento e ferro in stile liberty all'interno di un'aiuola alberata. Voglio inoltre precisare che il progetto attuale tende, per quanto possibile entro uno spazio a geometria fortemente irregolare, ad una ricomposizione degli elementi - alcuni di nuova concezione, ma comunque rievocativi della presenza del citato corso d'acqua tombinato - caratterizzanti la piazza, con un disegno suggerito dall'impostazione assolutamente simmetrica della facciata di palazzo Berzieri. Nel ridisegno del piazzale vi rientrano a far parte il Pozzo Scotti e l'aiuola attigua a cui ha fatto riferimento l'interrogante. Per quanto riguarda il Pozzo Scotti, il progetto propone una valorizzazione della visibilità e dell'ampia godibilità tutt'attorno al manufatto, mentre per l'aiuola (anche in considerazione del fatto che alcune essenze arboree soffrono di gravi patologie che mettono in serio pericolo l'incolumità delle persone) gli elaborati progettuali propongono una ricomposizione formale dettata dalla salvaguardia degli elementi arborei ancora sani e dalla soppressione, limitata ai soli esemplari malati di alcune essenze a medio e alto fusto. La presenza delle aiuole, rivisitate col progetto, non viene quindi né ridotta, né eliminata, ma compensata mediante il ridisegno delle aiuole laterali all'atrio d'ingresso delle terme e l'inserimento di un aggiuntivo spazio verde strettamente connesso al nuovo specchio d'acqua. Tali spazi verrebbero inoltre proposti come spazi ove sarà possibile praticare le attività di mosaicoltura. come già evidenziato, per il piazzale vuole essere rievocativo della presenza del torrente Citronia e dello stretto legame che sussiste fra quei territori padani e il proprio reticolo idrografico), di dimensioni contenute, posto sul bordo estremo dello slargo, non entra in conflitto con l'architettura delle terme, ma consente una delimitazione dello spazio antistante alle terme stesse, mitigando la presenza del traffico che transita dal viale attiguo ad esse. Sulla base di quanto esposto, faccio pertanto presente che il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso i suoi uffici territoriali, ha provveduto in data 29 giugno 2009

che i materiali previsti per la pavimentazione del piazzale e della fontana siano necessariamente sottoposti alla preventiva valutazione della locale soprintendenza, nonché l'assoluto divieto a modificare l'andamento altimetrico delle aree a colture a verde, onde evitare qualsiasi alterazione della percezione visiva dalla parte basamentale della facciata delle Terme Berzieri.

ha sicuramente rassicurato me, ma soprattutto i cittadini di Salsomaggiore, sull'attenzione da parte del Ministero per i beni e le attività

che lo stile del palazzo, che attinge i propri elementi e i propri motivi sia dal liberty che dal déco e che rende Salsomaggiore una città unica al mondo per la qualità e l'unicità dei suoi edifici, sia salvaguardato e sia sotto l'attenzione del Ministero e della sovrintendenza. Mi ha fatto poi particolarmente piacere sentire la sottolineatura che, nella scelta dei materiali che saranno utilizzati, questi saranno sottoposti alla valutazione della sovrintendenza locale. Voglio solo ricordare, in questa occasione,

dei medici, come Berzieri, e degli imprenditori del luogo, è diventata un luogo d'arte ma anche un luogo importante di salute e di cura.

viari e, quindi, destinati a divenire viali alberati e percorsi dell'architettura del verde. Voglio ricordare che Voglio ricordare che proprio una legge del Parlamento ha sancito il passaggio dell'industria estrattiva e termale dalla concessione ai privati alla gestione diretta del demanio. Con un provvedimento specifico, lo Stato finanziò la costruzione del nuovo grande stabilimento inaugurato nel 1923.

Questo significato aveva la mia interrogazione, al fine proprio di valorizzare splendidi monumenti del patrimonio nazionale